in questo breve intervento vorrei esprimere il rammarico per un'occasione perduta qual è questo provvedimento, e non soltanto perché questo ramo del Parlamento è stato privato sostanzialmente e formalmente della possibilità di incidere in modo significativo su di esso. Sappiamo bene che la tempistica strettissima della conversione del decreto lo rendeva di fatto inemendabile,

fatto inemendabile per i tempi di conversione, ma probabilmente lo è anche politicamente, visto che alla Camera,

la portata di un provvedimento di straordinaria incisività per contrastare la fortissima crisi economica che sta mettendo in grave difficoltà il Paese,

invece questo provvedimento manca al suo obiettivo fondamentale di rispondere con equità Quando ho preso atto della condizione di limitatezza assoluta che il Senato avrebbe avuto rispetto

tante iniziative emendative, tante interlocuzioni con gli amici del Governo, i relatori di maggioranza e i Presidenti di Commissione, che poi ogni volta deludono deludono le nostre aspettative. In questo caso, in fondo, questo rito mi era personalmente risparmiato, visto che era stato consumato alla Camera dai miei colleghi, che hanno prodotto iniziative parlamentari serie e rigorose, tutte perfettamente nell'alveo delle indicazioni del Governo, e che hanno trovato una risposta unica, immodificabile e ripetitiva sino all'ossessione: no, no, no. Non ci sono soldi, non c'è nessuna possibilità, non c'è alcuna praticabilità per le vostre iniziative emendative. Ma questo, signora Presidente, non toglie nulla...

questo tempo e assolto alla mia funzione di ricordare. Non smetterò infatti di ricordare al Governo e alla maggioranza parlamentare che in tutti gli atti che stanno affrontando i temi economici c'è un grande assente, il Sud, ma c'è anche un altro grande assente: il programma di Governo. Amici

perché il Sud del Paese gli ha tributato un consenso forse sproporzionato per l'attenzione che gli viene oggi riservata. Sapete cosa era riportato nel punto 5, che veniva prima del punto 6, sul federalismo fiscale? Si legge: «Noi vogliamo un'Italia che finalmente superi, attraverso un impegno straordinario, il drammatico divario tra Nord e Sud, realizzando una politica che valorizzi la responsabilità dei territori e metta a frutto tutte le energie presenti nel Paese». Sapete qual è la risposta di questo provvedimento? Il Governo prevede la possibilità di zonizzare le tariffe energetiche, differenziandone il costo e facendolo pesare

a imprese e famiglie. Ma vi rendete conto che questa è un'offesa all'intelligenza e all'equità? Io spero che almeno questo ordine del giorno approvato alla Camera...

io stesso. La scortesia che vi riservo, di farvi gravare questo tono così alterato, è quindi il frutto di una condizione ambientale anch'essa un po' inquinata dal rumore di fondo.

Vorrei esemplificare ulteriormente le nostre perplessità sul provvedimento. Non torno sul tema dell'utilizzo dei fondi FAS, perché si tratta di una tiritera che ormai ha stancato tutti, tranne chi ovviamente sente il peso di queste scelte. il Presidente del Senato metta all'ordine del giorno le mozioni sui FAS, che tutti ebbero cura di produrre dopo la mia iniziativa, compreso il Gruppo del PdL, che fu

Il Governo interviene giustamente per garantire stabilità alle banche perché occorre garantire i risparmiatori. Mi aspetto però che il mio Governo prenda in carico il tema della differenza inaccettabile tra il costo del denaro al Sud rispetto al Nord. Le nostre famiglie e le nostre imprese pagano di più il denaro, imprese pagano di più il denaro, perché le condizioni di difficoltà economiche e i rischi che esse assumono sono più gravi, e quindi le banche si garantiscono. Le nostre banche si sono industriate in derivati, in finanza creativa e i loro manager per qualche tempo sono stati *maître à penser* in questo Paese, titolari di un potere invasivo e qualche volta oscuro. Rispetto a tali manager, che spesso vengono salvaguardati nelle loro responsabilità, il Governo intervenga oltre la *moral suasion*,

altra preoccupazione. Adesso aleggia l'ipotesi che i fondi strutturali vengano utilizzati non soltanto per gli ammortizzatori sociali, termine generico ma sappiamo che cosa vuole dire. Tuttavia, noi al Sud abbiamo poco da essere ammortizzati, perché siamo già allo scontro frontale; gli ammortizzatori vanno da altre parti! Ciò vuol dire che i fondi strutturali, da aggiuntivi che dovevano essere rispetto agli ordinari,

alla Camera si può distinguere tra fiducia e voto sul merito del provvedimento. I miei colleghi l'hanno fatto: hanno votato la fiducia, ma non hanno votato il provvedimento. Questo Regolamento, che garantisce la funzionalità e l'agilità parlamentare ma garantisce anche molto il Governo, non me lo consente. Allora, come ho sempre ricordato, il mio voto di fiducia non mancherà perché il mio vincolo alla coalizione rimane intatto: è un voto neutro politicamente, doveroso, che risiede in un accordo politico preesistente.

a votare, è una fiducia che mi costa moltissimo.

anche in Conferenza dei Capigruppo, riteniamo che, se il Governo ha deciso di legiferare in via ordinaria attraverso decreti delegati e decreti-legge, venga in Parlamento a dirlo, così evitiamo di perdere tempo. Se il Senato e la Camera sono considerati un inutile orpello che allunga i tempi delle decisioni basta dirlo. Guardate, colleghi, noi siamo costretti a un voto di fiducia su un provvedimento che dovrebbe essere risolutivo dei problemi economici di tanti italiani,

Si è trovata, dunque, una mediazione interna alla maggioranza, codificando quella che era una prassi, vale a dire l'ampliamento delle concessioni in deroga per gli *slot* su Malpensa,

che doveva avere un valore strategico per lo sviluppo e il risanamento economico-finanziario del Paese e che in realtà si è trasformato nel punto di equilibrio e di tenuta della maggioranza di Governo.

con riferimento alla necessità di individuare una marcia in più per tutelare i soggetti deboli del nostro Paese, che non sono tutelati (con particolare riferimento alla famiglia)

cominciato con il federalismo fiscale, che sarebbe stata la leva per far cambiare tutte le politiche economico-finanziarie ed affrontare la crisi mondiale congiunturale. il federalismo fiscale, che - Dio non voglia! - si realizzerà tra sette anni, dovrebbe risolvere i problemi congiunturali della crisi economica che proviene dagli Stati Uniti. Siamo quindi passati ai 30.000 militari per le strade delle città, anche questi soldati del bene e, quindi, anche del bene economico.

pone in secondo piano l'esame impietoso della situazione economica e sociale di questo Paese e delle misure che sono necessarie per uscire dalla crisi. Questo è il dato politico che registriamo

delle politiche di risanamento dei conti pubblici del nostro Paese? Cito dati ISTAT che possono essere discussi, ma - mi auguro - non messi in discussione per la loro attendibilità: il livello di il livello di indebitamento del nostro sistema economico-finanziario pubblico, nei primi nove mesi del 2008, è pari al 2,1 per cento del prodotto interno lordo;

e una validità limitata solo all'esercizio 2009. Per quanto riguarda gli interventi sulle famiglie,

Sono dati accertati e certificati e sui quali non vi è alcuna possibilità di correzione neanche qui in Senato, considerato che è stata posta la fiducia. A ciò dobbiamo aggiungere che non vi è alcuna traccia, nemmeno tendenziale, di quelle politiche sul quoziente familiare di cui tanto qualcuno si riempie la bocca e che non si ritrovano, neanche per cenni, in questo provvedimento che dice di voler risollevare le sorti delle famiglie italiane meno abbienti.

nel capitale e nel patrimonio delle banche, sia funzionale alla tutela delle famiglie e delle imprese italiane. Signor Presidente, per queste ragioni riteniamo che il voto del nostro Gruppo parlamentare non possa che essere contrario alla fiducia. Riteniamo che di altro abbia bisogno questo Paese che non di un provvedimento che potremmo metaforicamente censurare in questi termini: la montagna ha partorito un topolino inutile che cerca di dare tutto a tutti e che non dà niente a nessuno, dilapidando quelle poche risorse che invece dovrebbero essere usate prioritariamente per le famiglie italiane.

questa è la valutazione e la sintesi oggettiva che noi dell'Italia dei Valori ci sentiamo di fare, sia sulla questione di fiducia posta oggi dal Governo sia sull'inconsistenza dei provvedimenti contenuti nel decreto-legge n. Le modalità con le quali si è giunti alla conclusione di questo *iter* parlamentare mettono in evidenza una grave debolezza della maggioranza e del Governo. della maggioranza perché, nonostante i numeri, al suo interno vi è un'insofferenza malcelata sulla condivisione delle priorità del Paese. Le divergenze più recenti sono emerse sulle questioni della giustizia e del federalismo, sulla questione dei tagli al Sud, per la quale l'MPA di Lombardo già alla Camera aveva minacciato di non volere votare la fiducia (mentre per noi la questione meridionale è questione prioritaria), sulla questione Malpensa, sulla questione immigrati, con Maroni che vuole la tassa sugli immigrati e il Governo che una debolezza del Governo perché la scelta del metodo della decretazione d'urgenza altro non è che il manifesto politico del nuovo corso del centrodestra, che è passato dal profilo identitario neoliberista del periodo 2001-2005, che ha causato danni evidenti in termini di deficit, di debito e di mancato controllo della spesa corrente (tant'è che alla fine di quella esperienza il Paese dovette rientrare da un'infrazione comunitaria per il 4,5 per cento a un profilo identitario improntato a un decisionismo autocratico e compassionevole, che creerà un danno non meno grave e pericoloso. Di ciò ha già preso coscienza la stessa Corte dei conti, nella sua relazione annuale alle leggi di spesa ha stigmatizzato che il ricorso eccessivo ai decreti non solo presenta profili di carattere ordinamentale, conseguenti all'indebolimento della partecipazione parlamentare alle decisioni di spesa, ma appare indubbio che all'approvazione delle leggi si pervenga a volte senza un adeguato approfondimento sulla congruità degli stanziamenti rispetto alle esigenze che si intendono soddisfare.

Egli si è limitato a ripetere che la profondità della crisi sta nelle nostre mani e che bisogna aver paura di avere troppa paura. Poiché sta nelle nostre mani e - aggiungerei - sulla pelle di tante famiglie e lavoratori, sul contenuto di questo decreto legge prevale da parte nostra una forte, seria e responsabile preoccupazione per le troppe assenze che vi ravvisiamo. Una prima grande assenza è la piena consapevolezza della crisi da parte del Governo. Il ministro Tremonti ci ha ricordato che l'Europa è in forte recessione, ma che l'Italia sta meglio. Non ci sentiamo eversivi se affermiamo che questa è una frase da campagna elettorale e non di chi vuole risolvere i problemi. I dati europei, che confermano quelli della Banca d'Italia, non sono congetture, ma lo scenario con cui chi ha responsabilità politiche deve misurarsi fino in fondo. Il circuito della fiducia non si attiva con la propaganda o nascondendo le cifre, ma proponendo e attuando politiche condivise che aggrediscono i punti di maggiore sofferenza, come la garanzia di un reddito per i nuovi disoccupati e il sostegno alle nuove povertà dilaganti. Purtroppo, il Governo non ha avuto né la capacità né il coraggio, nel decreto anticrisi, di dare risposte vere su nessuna di queste grandi questioni. Questo è ciò che fa male alle aspettative dell'economia, non le previsioni delle istituzioni preposte al monitoraggio. La preoccupazione che il peggio debba ancora arrivare, del resto, è presente in settori vitali e diffusi del nostro Paese. La stessa Confindustria, che ha avviato una pressione sul Governo per ottenere il potenziamento del decreto anticrisi varato a novembre, ha fornito nuove stime sullo stato di salute dell'economia nel prossimo futuro. La recessione nel 2009 sarà pesantissima, con una flessione dell'1,3 Per capirci, tra dodici mesi gli italiani avranno prodotto meno beni e servizi per oltre 24 miliardi di euro, con la perdita di oltre 600.000 posti di lavoro. Un'altra grande assenza, signor Presidente, è dunque una risposta adeguata in termini di tempestività, interventi mirati e politiche coordinate messe in campo dal Governo. Basta confrontarsi con il piano anticrisi definito a Bruxelles. Lo schema del provvedimento della Commissione europea prevede un coordinamento delle economie europee e dei rispettivi sforzi: 200 miliardi di euro di incentivo complessivo immediato, di cui 170 miliardi a carico degli Stati membri. Questo significa che lo sforzo maggiore dovrà essere a carico dei singoli Stati, Italia compresa. Così la Così la Germania ha presentato un piano di sostegno all'economia di 50 miliardi di euro, mentre il Governo britannico, solo per mitigare la stretta creditizia che colpisce le piccole e medie imprese, ha annunciato un intervento da 22 miliardi. L'ennesima grande assenza in questo decreto-legge è rappresentata dalle risorse economiche. La sommatoria di iniziative contenute nell'articolato del decreto non è nient'altro che l'uso di un contentino generalizzato e spalmato a pioggia al fine di conservare un consenso superficiale del Governo, che i sondaggi dicono essere a rischio, ma l'obiettivo è così scoperto e irresponsabile da far perdere fiducia anche ad associazioni di categoria che non si possono certo definire di sinistra. Il decreto anticrisi si limita, in pratica, ad una modesta redistribuzione di risorse in un gioco delle tre carte, perché la manovra si è andata sgonfiando nel tempo, la stessa comporta costi amministrativi sproporzionati in rapporto alle erogazioni e ai vantaggi realmente concessi ai cittadini e si crea tanta burocrazia, ma nessun posto di lavoro. Si è detto comunque che si tratta di una manovra a saldo zero (lo si è ripetuto anche in quest'Aula durante il dibattito), perché non peggiora i conti pubblici. In realtà il decreto anticrisi ha effetti molto diversi da quelli presentati dalla Ragioneria generale dello Stato, in quanto sono sovrastimati i maggiori introiti da accertamento e, soprattutto, esso consente lo smantellamento delle misure antievasione approvate nella scorsa legislatura, come la revisione in corso per via amministrativa degli studi di settore e l'introduzione di un paio di modifiche alle norme sull'accertamento. tra maggiori entrate inventate e perdite di gettito da evasione allargata, da giugno ad oggi la differenza tra manovre formali ed effettive è per il 2009 tra maggiori entrate inventate e perdite di gettito da evasione allargata, da giugno ad oggi la differenza tra manovre formali ed effettive è per il 2009 quasi un punto percentuale di PIL, a danno di lavoratori dipendenti, di pensionati e di precari, che ricevono solo qualche briciola attraverso la *social card*, il *bonus* famiglia e qualche sussidio disoccupazione in deroga.

un sistema di detrazioni fiscali legate realmente al numero dei componenti delle famiglie, una diversa distribuzione della ricchezza attraverso interventi di politica fiscale e provvedimenti strutturali sugli ammortizzatori sociali a maggior tutela del lavoro flessibile. Secondo l'analisi del centro di ricerche CERM, se si considera il *bonus* di importo massimo e la *social card*, saranno in pochissimi della già stretta platea di riferimento a beneficiare del tetto massimo, mentre se consideriamo il valore minimo più diffuso dell'*una tantum* e un valore intermedio per le agevolazioni tariffarie, si arriva ad un valore molto più contenuto, pari mediamente a 20-30 euro in più al mese. Questo è quello che mettiamo nelle tasche delle famiglie che hanno bisogno nel nostro Paese. Nel provvedimento una grande assenza è il disegno di un quadro strategico nazionale. La riduzione delle tasse non era l'obiettivo principale di questo Governo? Nel dibattito in corso su quali siano le misure per uscire prima dalla crisi e ritrovare la crescita, non sono pochi gli economisti che chiedono proprio i tagli alle tasse, sia per i privati sia per le imprese. Anche il Governatore della Banca d'Italia sostiene che per superare la crisi l'unica soluzione sia ridurre il peso del fisco, mentre la Gran Bretagna di Gordon Brown diminuisce l'IVA, Barack Obama annuncia tagli, Angela Merkel ha deciso di usare il bilancio dello Stato per contrastare la crisi. Noi in Italia, nel 2009, signor Presidente, dovremo lavorare due giorni in più rispetto al 2008 per pagare le tasse. Risulta dall'annuale statistica del *tax freedom day*, che calcola quanti giorni lavorativi sono necessari a un cittadino per far fronte agli impegni fiscali. Sono state confermate le decisioni contenute nel DPEF triennale per cui il carico fiscale rimarrà praticamente invariato fino al 2013, addirittura aumentando di due decimali nel 2010. Signor Presidente, in questo decreto-legge c'è un'unica grande presenza: la permanenza dell'attesa per i bisogni reali della gente. Il Paese ha bisogno di una politica forte e condivisa. Se deve prendere atto di verità amare sotto il profilo dei conti, ha un diritto in più per conoscere la verità dei fatti senza distorsioni mediatiche. Non sono parole nostre, dell'Italia dei Valori, ma è l'appello che il presidente della CEI, cardinale Bagnasco, ha rivolto oggi sulla stampa. Con il nostro voto convintamene contrario, con l'unica possibilità che ci è stata lasciata in questo Parlamento, a noi spetterà il compito e il dovere di far conoscere alla gente questa verità e fare in modo che, in futuro, i cittadini non debbano subirla. Grazie, Signor Presidente, colleghe e colleghi, la Lega Nord voterà la fiducia sul decreto anticrisi Nel merito, il provvedimento contiene una serie di interventi che la Lega valuta positivamente e condivide in pieno. Faccio qualche esempio: il noto emendamento salva-Malpensa sulla liberalizzazione delle rotte; gli interventi a favore delle imprese (soprattutto quelle più piccole); la revisione congiunturale degli studi di settore (anche se sappiamo che c'è da fare ancora di più su questo tema); l'IVA per cassa; il rimborso IVA soprattutto per le auto aziendali; la detassazione dei contratti di produttività e di innovazione; la deduzione dell'IRAP dall'IRES, almeno per il 10 l'importante intervento sui confidi, potenziati per 450 milioni; l'abolizione della commissione di massimo scoperto; e poi gli interventi di carattere sociale tra i quali il *bonus* per le famiglie in difficoltà, da 200 a 1.000 euro, e l'incremento degli assegni familiari.

Innanzi tutto, ricordiamo che, fortunatamente, abbiamo anticipato il grosso della manovra con il famoso decreto-legge n. 112, a luglio dello scorso anno. Il fatto che oggi si possa serenamente discutere di politica economica senza avere pesanti ripercussioni

L'effetto positivo di questa azione prudente del Governo si evidenzia con la tenuta del *rating* del nostro debito pubblico. Alcuni professoroni anglosassoni ci chiamano con un certo disprezzo "PIGS", parola che significa "maiali" ma che è anche l'acronimo di quattro Nazioni del Sud Europa: Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. Ebbene, solo la nostra Nazione, rispetto alle altre, ha tenuto sul *rating* del debito pubblico e questo è molto importante, perché ci consente di non avere pesanti effetti sull'incremento del costo del debito stesso. Se vogliamo, è una piccola rivincita del sistema nostrano, soprattutto padano, ma anche di altre parti d'Italia, di quel sistema di piccole e medie imprese, rispetto a una visione così, che andava di moda, *post*-industriale; è la rivincita dell'economia reale sull'economia finanziaria e globalizzata. presto però per cantare vittoria. Per ora stiamo tenendo molto meglio di tante Nazioni europee. Il rapporto *deficit-*PIL sarà, a fine anno, del 3,8 per cento, molto meglio di altre Nazioni, quali Francia, Spagna, Irlanda e Inghilterra. Perché stiamo tenendo meglio? Quali sono i nostri punti di forza attuali, su cui lavorare ancora e meglio in futuro? Soprattutto il tessuto diffuso di piccole, piccolissime e medie imprese, artigiani, commercianti; l'economia reale, manifatturiera, insomma. Poi il sistema, anche questo diffuso e molto legato al territorio, di banche popolari e cooperative, le stesse che fino a qualche mese fa erano sotto tiro perché si diceva che erano troppo piccole e bisognava inglobarle nelle grandi banche, che poi hanno fatto i disastri che abbiamo visto. E ancora,

Purtroppo, però, questa propensione al risparmio sta calando in maniera molto preoccupante e anche su questo occorrerà intervenire. La Lega Nord, quindi, chiede che nei prossimi interventi di politica economica, che - siamo certi - ci dovranno essere per forza visto l'evolversi della crisi economica mondiale, si agisca proprio su questi che sono i nostri punti di forza. forza. Ad esempio, noi chiediamo interventi per dare davvero liquidità al sistema delle piccole e medie imprese. Le banche non chiedono i soldi che lo Stato ha messo a disposizione: bisogna fare qualcosa affinché ciò avvenga, affinché torni liquidità al sistema delle piccole e medie imprese. Chiediamo poi la revisione certa, effettiva, degli studi di settore. Si dice sempre che gli studi di settore sono una statistica: ebbene, se lo sono e non sono una *minimum* *tax*, perché perché non applicare la presunzione semplice? Infine, ancora ad esempio, chiediamo la modifica dal Patto di stabilità interno, soprattutto per i Comuni virtuosi. Noi proponiamo che per i Comuni virtuosi, per la spesa di investimento, si liberi la possibilità di spendere quattrini. Questo è un altro modo per dare subito fiato all'economia, anche perché le asfaltature non si possono importare e ciò costituirebbe davvero un aiuto reale e concreto al nostro sistema produttivo. In conclusione, signor Presidente e colleghi, una nota di ottimismo: paradossalmente abbiamo un'enorme possibilità che ci viene proprio dalla spesa pubblica, abnorme e fuori controllo. Il fatto di avere una spesa pubblica superiore al 50 per cento del PIL, cioè del fatturato totale del sistema Italia, ci consente enormi margini di miglioramento. Rispetto ad altre Nazioni che hanno uno Stato snello possiamo agire con tagli mirati alla spesa pubblica; non più i tagli lineari degli anni scorsi, che poi si traducono in necessarie reintroduzioni di spesa, ma tagli mirati dove ci sono sprechi. Per dare l'idea, un solo taglio del 5 per cento di quei quasi 800 miliardi di euro di spesa pubblica vale ben 40 miliardi di euro l'anno, tutti gli anni. 40 miliardi di euro sono quattro finanziarie; 40 miliardi di euro è la metà del costo del debito pubblico, la metà degli interessi che paghiamo sul debito pubblico. Non diteci che è impossibile tagliare la spesa pubblica del 5 per cento: ogni cittadino uscendo dalla propria abitazione può vedere quali e quanti sprechi ancora ci sono nel sistema pubblico italiano. Ebbene, la Lega Nord da tempo ha indicato come effettuare il taglio della spesa pubblica; la soluzione c'è ed è alla nostra portata: si chiama federalismo e, in particolare, federalismo fiscale.

che oggi siamo chiamati a convertire con il ricorso al voto di fiducia, per l'undicesima volta nei due rami del Parlamento in otto mesi di legislatura, è il trentaquattresimo, a fronte dei 19 dello stesso periodo della precedente legislatura, pur in condizioni, politiche e numeriche, di sostenibilità del lavoro parlamentare enormemente differenti ed a fronte dell'inesistente ricorso da parte nostra a qualsiasi strumento di ostruzionismo o di ostacolo all'attività parlamentare (per questo provvedimento non abbiamo neanche presentato questioni pregiudiziali e sospensive). Si tratta, come abbiamo già avuto modo di denunciare più volte, di una scelta politica senza precedenti, che sta producendo un mutamento sostanziale della Costituzione materiale del nostro Paese, tutto a favore di un Governo ostile a qualunque virtuoso confronto parlamentare e tutto a danno delle Assemblee legislative rappresentative della volontà popolare. A nulla sono valsi fino ad oggi i richiami delle più alte cariche dello Stato e delle opposizioni al recupero della centralità del Parlamento sulla base della lettera e dello spirito democratico Il Governo continua a marciare su un binario di prevaricazione della dialettica democratica, la maggioranza è silente e ratifica, le opposizioni propongono misure alternative e migliorative dei testi dei testi legislativi senza incontrare attenzione e ascolto nella quasi totalità dei casi, con l'unica eccezione positiva del federalismo fiscale. Tale lesione delle prerogative del Parlamento ha assunto il carattere della patologia grave qui al Senato della Repubblica. Quasi tutti i provvedimenti contenenti misure economico-finanziarie, recanti interventi lordi per circa 49 miliardi di euro, in otto mesi, in gran parte costituiti da tagli alle spese, sono stati approvati o con la fiducia o senza modifiche. Il numero degli emendamenti approvati si conta sulle dita di una mano ed essi hanno inciso, in misura marginalissima, solo su due provvedimenti. Tale dato politico, al quale non intendiamo rassegnarci, assume una connotazione ancor più inaccettabile a fronte della gravissima crisi economica che è in atto, la più lunga e pesante dal dopoguerra. In tutti i Parlamenti delle Nazioni democratiche, i Governi, le maggioranze e le opposizioni si confrontano, cooperano per la ricerca della migliore soluzione per fronteggiare e uscire dalla crisi. In Italia, invece, ciò non è possibile. I Capi dei Governi e i Ministri dell'economia vanno nei Parlamenti e spiegano le strategie e le misure necessarie. Noi qui non abbiamo né visto né sentito il Presidente del Consiglio, né il Ministro dell'economia e delle finanze, in Aula. In Italia ciò non è possibile non perché l'opposizione non è disponibile o perché gioca al «tanto peggio, tanto meglio»! No, non è possibile per scelta politica del Governo e della maggioranza che irresponsabilmente non ascoltano, rifiutano il confronto, non si fanno carico di suscitare uno spirito di cooperazione nazionale per affrontare il dramma di milioni di famiglie, la crisi del sistema delle imprese, le enormi difficoltà dei conti pubblici. Noi abbiamo detto e ribadiamo che siamo disponibili a dare il nostro contributo. Abbiamo formulato proposte precise, coperte finanziariamente, ispirate non da una logica di contrapposizione ma dal convincimento profondo che altro servirebbe oggi al Paese per mostrarsi all'altezza della grande sfida che la crisi ci obbliga ad affrontare, per superare l'emergenza e per immaginare oggi come sarà il Paese dopo la crisi. Nel mondo, nelle altre Nazioni a noi più vicine per struttura economica e sociale, non soltanto l'ispirazione politica di costruzione di una risposta alla crisi è molto diversa dalla nostra, ma la qualità e la quantità degli interventi attuati, messi in cantiere o annunciati sono enormemente superiori a quelli sin qui partoriti dal vostro Governo: 73 miliardi in Germania, 41 miliardi in Spagna, 26 nel Regno Unito; 825 miliardi di dollari negli Stati Uniti d'America di Barack Obama, da investire nell'ambiente, nelle energie alternative, nell'istruzione, nelle infrastrutture, nel *welfare*, i pilastri di ciò che sarà quel Paese dopo la crisi. E noi? Una manovretta da 5 miliardi di euro, con un impatto stimato sul PIL di un decimo di punto, con interventi *una tantum* o contrastanti con le necessità dell'oggi e del futuro. Un'occasione perduta, come l'ha definita poco fa il senatore Pistorio, che fino a prova contraria fa parte della maggioranza di Governo. Il Paese vedrà cadere il PIL del 2,1 per cento nel 2009, come ci dicono l'Unione europea e il Fondo monetario internazionale? Ma non è mica il ritorno al Medioevo, dice il ministro Tremonti! Ignorando o facendo finta di ignorare che dietro quel dato medio ci saranno nei prossimi mesi, e non lo diciamo noi ma Confindustria, 600.000 posti di lavoro in meno, l'esplosione della cassa integrazione, cento in più di disoccupazione, il raddoppio dei fallimenti delle aziende, il 13 per cento in meno di produzione industriale, il 10 per cento in meno di investimenti fissi in attrezzature, il 17 per cento in meno di investimenti pubblici in meno e così via. Il settore dell'automotive, non solo la FIAT, è investito da una gravissima crisi? Le previsioni nere rese note oggi ci dicono che per il 2009 ci sarà una riduzione del 60 per cento delle vendite e 60.000 posti di lavoro a rischio? Il ministro Calderoli, qui presente, dice: in caso di aiuto alla FIAT ci sarà una rivolta di popolo! Il mondo accelera e investe sulle energie alternative, sulla riqualificazione energetica degli edifici, sulle auto ecologiche per abbattere la dipendenza dal petrolio, sull'abbattimento dei gas serra anche per creare nuovi posti di lavoro? Noi non facciamo nulla e l'unico intervento è quello dell'indebolimento del principale e più efficace strumento messo in campo dal Governo Prodi, la detrazione automatica del 55 per cento per il recupero degli edifici in funzione del risparmio energetico che stava funzionando, eccome! La povertà in Italia aumenta? Il 13 per cento della popolazione vive con meno di 500-600 euro al mese e milioni di famiglie sono a rischio di povertà o hanno visto drasticamente ridurre il loro livello di reddito? In Italia, si inventa la macchinosa e caritatevole *social card* per poche persone, non si fa assolutamente nulla per accrescere i redditi di milioni di persone che non ce la fanno e si divide il sindacato nell'accordo per la riforma della contrattazione collettiva. Potrei continuare, ma non lo faccio per ragioni di brevità. L'unica risposta del Governo e del Ministro dell'economia è: abbiamo il terzo debito pubblico al mondo (lo abbiamo ascoltato anche oggi qui), abbiamo scelto di stabilizzare la finanza pubblica in anticipo, a luglio, non si può fare di più, non ci sono le risorse. La nostra parte politica era ed è per il rispetto dei vincoli di bilancio e del patto con l'Europa. Abbiamo dato ampia dimostrazione su questo rimediando ai danni degli anni della vostra finanza allegra e creativa e riducendo deficit e debito. e debito. Abbiamo anche pagato un enorme prezzo politico per essere stati coerenti e rispettosi delle regole. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ma limitarsi alla constatazione ovvia dei vincoli di finanza pubblica significa condannare il Paese all'immobilismo, significa non avere, come voi non avete, una politica anticrisi. Potremmo, sul punto, limitarci a ricordarvi che avete intenzionalmente dissipato nei mesi scorsi 7-8 miliardi di euro per provvedimenti sbagliati quali quelli su ICI e Alitalia, che avete colpevolmente depotenziato gli strumenti di lotta all'evasione fiscale che stava dando

Grazie, sistema di ammortizzatori sociali universale che estenda le tutele reddituali a tutti, anche ai precari, misure per l'energia, per le infrastrutture e in particolare per gli investimenti degli enti locali, rivedendo le regole del Patto di stabilità interno come chiedono insistentemente i Comuni e anche qualche forza di maggioranza. Mobilitare un punto di PIL (questo abbiamo detto), almeno di 15 miliardi di euro nel 2009, con contestuale previsione di rientro attraverso misure certe di riduzione della spesa da adottare appunto contestualmente, con efficacia nel 2010 e nel 2011. Oppure, ulteriori interventi selettivi sulla composizione della spesa pubblica anche con interventi di riforma concordati ed immediati, per orientare la spesa verso ciò che serve, ovvero più giustizia sociale, più consumi, più investimenti e quindi impulso alla ripresa dell'economia. Nulla di tutto ciò viene viene da voi in concreto preso in considerazione e non è difficile prevedere che cosa accadrà nel prossimo futuro. Il deficit (già oggi risalito dal 2,3 per cento dell'aprile 2008 al 3,8 per cento) (passato dal 103,2 per cento dell'aprile 2008 al 109,3 per cento di oggi) peggioreranno ancora. La vostra politica economica restrittiva non potrà incidere sull'andamento dell'economia e l'assenza di una politica industriale renderà, come già sta accadendo, meno competitivo il nostro sistema II Paese si sta già accorgendo e si accorgerà ancora di più nei prossimi mesi che la vostra politica economica e di bilancio non risolve nulla e ci restituirà un Paese più ingiusto, più povero, meno competitivo e più indebitato. Potremmo rallegrarci per questa vostra conclamata incapacità ad affrontare la crisi ma non vogliamo farlo perché sarà il Paese, i cittadini e le imprese italiane, a pagare il conto del vostro immobilismo. Noi non vogliamo arrenderci: si può e si deve fare di più. «Dalla crisi deve e può uscire una Italia migliore» e ciò sarà possibile se riusciremo "ad unire tutte le forze, a valorizzare le energie vitali, a superare le debolezze, a risolvere di slancio i problemi che ci trasciniamo": questo disse a noi tutti

ma sarete costretti dagli eventi a riconoscere - speriamo non quando sarà troppo tardi - i vostri errori e le vostre omissioni. signor Presidente, e per tutti quelli che i nostri colleghi hanno illustrato nei loro interventi, che il Gruppo del Partito Democratico negherà la fiducia al Governo. Signor Presidente, colleghi, sul piano procedurale non mi attarderò molto, perché so bene di non poter reggere in nessun caso il confronto con il precedente Governo Prodi:

Ripeto, certamente funziona in maniera incomparabilmente migliore della precedente legislatura, ma non è il caso appunto di soffermarsi a lungo su questo terreno,

Non ci si può dimenticare che questo decreto‑legge va inserito nel contesto di una manovra, che riteniamo equilibrata, efficace e preveggente, posta in essere dal Non va dimenticato che questa manovra comincia con l'anticipo a luglio della manovra triennale, che è stato determinante perché l'economia italiana reggesse nel miglior modo possibile allo scatenarsi della crisi che tutti conosciamo. E non solo. È stata determinante in uno degli aspetti più deboli della nostra situazione, quella del debito pubblico. Avremmo potuto avere una finanza pubblica fuori controllo nel corso di una crisi di questo tipo, e questo sarebbe stato rovinoso per l'Italia. La preveggenza del nostro Governo ha fatto sì che con la manovra triennale di luglio l'Italia, il debito pubblico italiano, la finanza pubblica italiana hanno potuto reggere alla crisi; tant'è che la stessa Commissione europea si è sforzata più volte di dire che, tutto sommato, di fronte a questo stravolgimento economico-finanziario, l'economia e la finanza pubblica italiana hanno retto meglio di altre. Ma non solo. La manovra di questo Governo ha trovato modo di attuarsi anche attraverso i decreti di fine anno, che hanno consentito

Ed anche lì è stato efficace il nostro modo di essere, un modo di essere non invasivo delle banche, ma pronto a dare una sponda molto seria ed efficace ad eventuali crisi di liquidità. Anche su questo la nostra manovra è stata così efficace che le banche, allo stato, non hanno ancora attinto alle garanzie, alle obbligazioni del Tesoro, ma quella

Ma ricordo a tutti, in particolare ai colleghi dell'opposizione, che lo sviluppo in Italia ha necessità, prima di tutto, di avere sotto controllo la finanza pubblica una deriva sotto quel profilo, nessuna misura di sviluppo potrebbe avere efficacia. Questo è il punto di sintesi del decreto-legge Voglio infatti sottolineare che sul piano quantitativo la manovra non è secondaria per il nostro Paese. È una manovra che cifra in dieci miliardi nel triennio, ma che cifra per la metà della somma, cinque miliardi, esattamente nel 2009.

del deterioramento dovuto alla riduzione notevole del tasso di crescita del PIL. Se ad una riduzione prevedibile delle entrate si fosse aggiunto un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, avremmo nuovamente avuto effetti rovinosi per la finanza pubblica. Sanno bene i colleghi che in questo momento, mentre noi discutiamo qui, le aste dei nostri titoli di Stato hanno un ottimo accoglimento sul piano della quantità, ma lo *spread* sul *Bund* decennale tedesco, che è l'indicatore della tenuta della finanza pubblica, registra ancora un peggioramento da parte dei titoli italiani; il che significa che bene facciamo a non peggiorare i saldi e a porre in essere manovre che si tengano

sono possibili perché, dopo quelle manovre di notevole entità, il loro debito pubblico è ancora largamente inferiore al nostro,

famiglie, i pensionati e i non autosufficienti, determinato in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo. La manovra si sforza quindi di avere carattere sociale, di essere di aiuto ai redditi più bassi e, insieme, di natura economica per tentare di aumentare i consumi.

Voglio ricordare, colleghi dell'opposizione, che l'IRAP sul costo del lavoro è stata una di quelle sciagurate misure di appesantimento del costo del lavoro che ha frenato lo sviluppo in Italia.

Altrettanto importante è l'introduzione dell'IVA per cassa, che rappresenta un tentativo serio di portare sollievo, non soltanto al conto economico delle imprese, ma anche al loro conto finanziario, perché in questo momento, com'è noto, le imprese hanno bisogno di liquidità. La fase di crisi della liquidità si è infatti spostata dalle banche alle imprese e con questo provvedimento noi ci poniamo il problema di farvi fronte e ritengo che lo facciamo in maniera efficace. efficace sarà la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per i lavoratori autonomi e per le piccole imprese, che costituisce una maniera seria e corretta di affrontare il problema delle piccole e medie imprese. In materia di lavoro viene prevista la fruizione di ulteriori strumenti a tutela del reddito in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro, con una concessione di ammortizzatori sociali in deroga. Non so se il Governo sta già approntando nuove misure in questo senso, ma certamente il problema degli ammortizzatori sociali e delle misure per la disoccupazione e la sospensione dal lavoro è ben presente

della finanza pubblica. Viene inoltre prorogato al 2009 il regime delle agevolazioni fiscali per i lavoratori del settore privato sulla parte di retribuzione legata ad incrementi di produttività (quella cosiddetta di secondo livello): si tratta di un tentativo di migliorare tutta la contrattazione per dare, insieme al lavoro, meno precarietà e più flessibilità. Questo è quanto il Governo sta tentando di fare, eliminando uno degli esempi classici che venivano dalla sinistra:

(uno di 60 milioni di euro a partire dal 2009 e l'altro di 150 milioni di euro a decorrere dal 2010), oltre al Fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie

nella sua agenda per fronteggiare questa crisi con misure efficaci è giornaliero e inserito in un quadro strutturale. Per questo voteremo convinti la fiducia su questo decreto-legge e al nostro Governo.

Benedetti Valentini, Berselli,

Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri,

Filippi Marco, Finocchiaro,

Marini, Marino Ignazio,

voti).* Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1315, di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: